La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 23 novembre. 23 novembre. Sulle mozioni relative alla Conferenza di Nairobi, all'ordine del giorno di oggi pomeriggio, i Gruppi avranno a disposizione quindici minuti ciascuno, anziché dieci come precedentemente stabilito. Subito dopo si passerà alla discussione del decreto-legge sulla pubblica sicurezza. La giornata di domani e, se necessario, la seduta antimeridiana di giovedì saranno essenzialmente dedicate all'esame del decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania e, in relazione ai tempi disponibili, al seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma degli esami di maturità. Il calendario di questa settimana è integrato con la votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni reiterate dalla senatrice Magnolfi, che avrà luogo a fine seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 novembre. Nella seduta antimeridiana di giovedì 9 novembre inizierà l'esame del disegno di legge comunitaria, che proseguirà la settimana successiva. A partire da giovedì 16 novembre, con prosieguo e conclusione nella settimana seguente, sarà discusso il decreto-legge collegato alla manovra finanziaria, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Sull'emergenza criminalità a Napoli, il Ministro dell'interno riferirà alla 1a Commissione permanente alle ore 14,30 di giovedì 9 novembre. Ove possibile, in relazione ai propri impegni internazionali, il Ministro degli affari esteri potrebbe rispondere al *question time* sui diritti umani in Cina nella seduta pomeridiana di giovedì 16 novembre. Ulteriori richieste avanzate dai Capigruppo saranno esaminate nella prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che sarà convocata nella mattinata di martedì 14 novembre. Presidente, capisco che il Governo abbia una vocazione mondialista

All'inizio del Novecento, quando la questione napoletana esplose, ci si confrontò in Parlamento su un progetto di piano di sviluppo della città

su Napoli e sui progetti di sviluppo. Non c'è nessun nesso con il decreto-legge per l'emergenza, che ha i suoi tempi e che va votato, in quanto è un problema antico, nel cui merito entreremo domani. Aggiungo, però, ma solo in positivo, che altro è discutere dell'emergenza Napoli, altro è discutere di quella Napoli che, vent'anni fa (ha ragione il senatore Novi),

Presidente, leggiamo sulla stampa di oggi che dalle audizioni e dalle osservazioni fatte sulla manovra finanziaria

Ora, vorremmo sapere, in riferimento a quanto dichiarato dal Governo in tutte le audizioni, nella Nota di aggiornamento, nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto fiscale in discussione in questo ramo del Parlamento e nella finanziaria all'esame dell'altro ramo del Parlamento, cosa sia successo. Intendiamo a punto fare alcuni rilievi rispetto alle osservazioni che in questo ramo del Parlamento sono state pronunciate in ordine agli effetti della sentenza sull'IVA. La circostanza che il Governo faccia delle dichiarazioni in sede comunitaria e non risponda alle richieste che vengono avanzate nei due rami del Parlamento e che le stesse vengano riportate da "La Stampa", "la Repubblica" e altri giornali

il Presidente del Consiglio e con il ministro Padoa-Schioppa e non - per quanto di gratificante esperienza, perché sono diventati Sottosegretari - con professori universitari. Vogliamo che la politica ritorni al centro del Paese. Vogliamo che il Presidente del Senato chieda al Ministro di venire finalmente in questa Aula. Senatore Ferrara, essere professore universitario comporta anche una certa preparazione; quindi, non mi pare una categoria da sottovalutare.

ci mettano in condizione di chiarire il punto specifico che il senatore Ferrara ha posto, in modo che possa riferire un rappresentante del Governo che segue direttamente il problema. Credo che sia una necessità perché quella posta dal senatore Ferrara è una domanda che merita una risposta; quindi pregherei, in giornata, di essere messi in condizione di poter dare una risposta.

signor Presidente. Signor Ministro, signora Vice ministro e rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, con l'esame del provvedimento che contiene disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché una delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, l'Assemblea del Senato della Repubblica è chiamata oggi a rivolgere la propria attenzione agli studenti del nostro Paese, agli adolescenti e ai ragazzi che crescono nella nostra società, lasciatemi dire, alla bellezza, allo slancio della loro vita, alla loro crescente responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo. Saluto gli studenti che stamattina stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna. Anche l'esame di Stato è un passaggio al futuro. E l'Italia oggi è impegnata soprattutto in questo: ad aprire vie alle nuove generazioni. anni, al termine della scuola superiore, quando una fase della loro vita si conclude e un'altra si apre, gli studenti hanno il diritto di veder valorizzata la propria esperienza scolastica e la Repubblica ha il dovere di accertare e dichiarare i risultati acquisiti: un passaggio della vita che è insieme personale e pubblico, un passaggio serio, di cui siano percepiti il rigore, la dignità, la trasparenza, il valore; un passaggio rispetto al quale il futuro - e cioè l'università, gli istituti della formazione tecnica superiore, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni e il lavoro il lavoro - non sia un obiettivo lontano, ma una prospettiva già presente nell'orientamento e nel raccordo con la fase terminale dell'istruzione secondaria, nonché nella valorizzazione dell'eccellenza. *(Brusìo)*. PRESIDENTE. Senatore Ladu, è proprio dietro la relatrice, la prego. Poi ci sono le tribune con una presenza forte di giovani studenti, che saluto a nome dell'Aula. *(Generali L'esame di Stato, dunque, dentro la vita dello studente, dentro la vita del Paese. Questa è la cifra del provvedimento in esame, volto a cambiare una situazione non più sostenibile che, secondo l'opinione comune, ha visto progressivamente venir meno il significato e l'autorevolezza dell'esame di Stato. Qui c'è una svolta, nella considerazione di una prescrizione prevista dalla stessa Costituzione, che all'articolo 33 colloca l'esame di Stato conclusivo nel contesto dei punti fondamentali dell'istruzione, là dove si parla della libertà di insegnamento, del compito della Repubblica nel dettare le norme generali e nell'istituire scuole statali, della parità scolastica, dell'autonomia ordinamentale, delle università, accademie, istituzioni di alta cultura. Siamo all'inizio della legislatura e sentiamo di dover rispondere ad un interrogativo: perché si comincia dagli esami di Stato, mentre ancora incerta è la definizione dell'istruzione secondaria superiore, nel passaggio da una legislatura all'altra? Risponderò così: per due ragioni. In primo luogo, noi non faremo la riforma di sistema. Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo ciò che va raddrizzato ed adegueremo ciò che va adeguato. Questo è il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle famiglie e al Paese. In secondo luogo, l'investimento sull'esame conclusivo prefigura la strategia, l'approccio e la prospettiva.

Prego quindi l'Aula di moderare quantomeno il brusìo. Prego, senatrice Soliani. SOLIANI, *relatrice*. Nella vicenda parlamentare dell'ultimo decennio, questa è la terza legislatura che inizia con un intervento sugli esami di Stato. Così avvenne nel 1997, con la legge n. 425, ripresa in questo provvedimento; così avvenne nel 2001, con la legge finanziaria, che modificò la composizione delle commissioni. Così avviene ora, con l'equilibrio e la misura che sono richiesti dalla materia e dai tempi dell'entrata in vigore rispetto alla vita della scuola, con la consapevolezza che intervenire su questo punto significa delineare una strategia: quello che avviene prima e quello che avverrà dopo sono già considerati qui, nell'esame di Stato. Dunque, si può partire dall'esame di Stato. Abbiamo su questo un precedente illustre. Richiamerò le parole di Benedetto Croce che, nella sessione 1919-1920, alla Camera dei deputati, presentò appunto un disegno di legge per la riforma degli esami che si esprimeva così, tre anni prima della riforma Gentile, forse rispondendo alla stessa domanda: perché cominciare dagli esami di Stato? Diceva Croce: «E poiché gli esami, consistendo essenzialmente in una funzione statale di riscontro dell'opera della scuola, non possono fare a meno di informare di sé e quasi di predisporre quest'opera, ognun vede che dalle norme d'esame, con le quali si determina l'obiettivo finale a cui la scuola deve tendere, questa desume anche le sue direttive». Ecco: dalla fine, dunque, si desume il principio. Dall'esame, la scuola. Il testo che oggi giunge in Aula è il n. 960, predisposto dal Governo e modificato nella 7a Commissione nel merito. In 7a Commissione abbiamo esaminato contestualmente i disegni di legge di iniziativa dei senatori Valditara ed altri, nonché Schifani e Asciutti, a riprova del valore della materia in esame, abbiamo svolto numerose audizioni (circa trenta) che hanno arricchito il nostro dibattito. Sono lieta di poter riferire all'Aula i risultati di un confronto aperto e costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo, che ha portato a migliorare e ad arricchire in diversi punti, alcuni dei quali assai significativi, il testo del Governo, come è bene che avvenga in una democrazia matura: un confronto che ha portato tutto il Parlamento ad una prima, seria riflessione sulla scuola in questa legislatura, in attesa di altre scelte impegnative. Questa riflessione ha portato a convergenze importanti sulla serietà degli studi per la formazione dei ragazzi italiani, sul valore pubblico del sistema di istruzione, costituito di scuole statali e non statali, sulla continuità dell'apprendimento negli anni precedenti la conclusione degli studi e negli anni successivi. Sono rimasti alcuni punti di divergenza in rapporto, ad esempio, alle scuole paritarie. Ringrazio dunque tutti i colleghi, ma in modo particolare i senatori Asciutti, Valditara, Marconi, Davico, Capelli, Pellegatta, Carloni, oltre che il vice ministro Mariangela Bastico e, naturalmente, la presidente Vittoria Franco. Richiamo, in particolare, il contributo dell'opposizione, segnatamente del Gruppo di Alleanza Nazionale, per il tramite del senatore Valditara, sul profilo di serietà culturale dell'esame, sul ruolo dell'Invalsi, sulla composizione delle commissioni, sull'autonomia dell'università. Richiamo altresì il contributo del Gruppo di Forza Italia, e del suo capogruppo senatore Asciutti, sulla serietà del percorso dei cosiddetti «ottisti», sull'INVALSI, sui crediti anche professionali che si possono riconoscere ai candidati esterni, sull'abbinamento delle commissioni degli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati. Richiamo inoltre il contributo del Gruppo Unione dei Democraticicristiani e di Centro, per il tramite del senatore Marconi, sulla serietà culturale dell'esame, sul colloquio e la sua valutazione, sull'importanza della delegificazione. Richiamo infine il contributo del Gruppo della Lega Nord Padania, per il tramite del senatore Davico, sulla nomina dei presidenti, sulla composizione delle commissioni, sulla lingua d'insegnamento, sulla terza prova, sulla valutazione e sull'orientamento. Signor Presidente, sull'asse rappresentato dal disegno di legge n. 960 vi sono stati pochi, essenziali emendamenti del Governo e della relatrice che hanno raccolto gli stimoli del dibattito e delle diverse proposte emendative. Importanti sono stati i contributi dei colleghi della maggioranza. Richiamo, in particolare, quello della senatrice Capelli del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, sulla composizione delle commissioni, sulla terza prova e sul punteggio; il contributo della senatrice Pellegatta del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani sulla valorizzazione delle materie tecnico-scientifiche, sull'orientamento e il raccordo con l'università, la formazione tecnica superiore, l'alta formazione artistica e musicale; il contributo della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti contro la dispersione scolastica e, insieme con la presidente Vittoria Franco, sulla necessità di potenziare le conoscenze tecnico-scientifiche. Colleghi, a mio parere tre sono i punti qualificanti del presente provvedimento: il primo è la natura pubblica dell'esame e il contrasto dei diplomifici, la serietà delle prove e dell'impianto, il valore del titolo di studio; secondo è la responsabilizzazione degli studenti e delle istituzioni scolastiche anche in ordine alla verifica dei risultati, nella valorizzazione dell'autonomia delle scuole;

coerenza interna e apertura all'esterno, esattamente come si configura oggi l'impegno dell'Italia verso se stessa e il suo domani. Questi punti sono rintracciabili nelle articolazioni del disegno di legge: l'articolo 1, relativo alla commissione all'ammissione degli studenti alle sedi d'esame; l'articolo 2, che introduce per la prima volta una delega al Governo in materia di orientamento e l'articolo 3, infine, che concerne disposizioni transitorie, finali e finanziarie e le abrogazioni. Dirò per sommi capi che all'esame di Stato vengono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti negli anni precedenti. Come si vede, qui c'è la richiesta del Parlamento rivolta alla scuola e agli studenti di un impegno più cogente. Possono poi accedere agli esami gli alunni che abbiano ottenuto nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascun disciplina e non meno di sette nei due anni antecedenti il penultimo. Inoltre, i candidati esterni possono sostenere l'esame di Stato presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel Comune di residenza. In questo passaggio, colleghi, vi è, da un lato, la coerenza con il profilo del sistema pubblico di istruzione costituito di scuole statali e scuole paritarie in relazione alla legge n. 62 del 2000 e dall'altro il contrasto ai diplomifici. A questo riguardo, desidero rilevare come complessivamente il disegno che giunge in Aula sia coerente con l'impostazione che al tema della parità scolastica hanno dato innanzitutto la Costituzione e poi la stessa

Italiani). Ebbene, l'Ulivo, il Gruppo Per le Autonomie e il Governo hanno difeso il baricentro rappresentato dal testo governativo. Il rispetto del ruolo pubblico delle scuole non statali paritarie implica che esse siano in condizione di parità con le scuole statali ma non sono previste, allo stato, condizioni di reciprocità per la presenza dei presidenti e dei commissari esterni, in ragione del ruolo e della funzione stabiliti per i docenti statali nelle commissioni, appunto, degli esami di Stato. Un ordine del giorno approvato in Commissione invita tuttavia alla formazione comune dei docenti e ciò è indicativo della volontà di qualificare tutto il sistema pubblico di istruzione.

per esempio, i ragazzi che hanno dato ottima prova del loro apprendimento possono anche conseguire la lode nel punteggio finale. Inoltre, sulla terza prova, affidata all'autonomia scolastica, è bene che si valutino i risultati dell'insieme delle prove con il contributo dell'INVALSI che offre modelli e contributi per il lavoro delle commissioni, ma con l'autonomia delle commissioni di esame, in grado, tuttavia, di rendere i risultati della scuola italiana comparabili con la valutazione internazionale. Cito infine la novità strategica di cui all'articolo 2: si investe sulla continuità dell'apprendimento negli anni decisivi della formazione e per tutta la vita, come avviene in Europa e nel resto del mondo sviluppato. Emerge dunque il profilo di una scuola seria, solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, che valorizza i talenti, che è attenta ai risultati, nell'interesse degli studenti italiani e nell'interesse del Paese; una scuola più europea. Presidente, mi avvio a concludere. Onorevoli colleghi, per le ragioni che ho esposto è bene non accumulare ritardi sulla vita degli studenti e sul Paese, che ne registrano già parecchi. È bene che il provvedimento sia approvato dal Parlamento ora, perché le istituzioni scolastiche possano prepararsi al nuovo esame fin da ora, a partire da questo anno scolastico. Non sarebbe opportuno rinviare l'applicazione delle nuove norme, come da qualche parte si sollecita, perché è bene fare presto ciò che può migliorare la vita della scuola italiana. Altri problemi relativi ai percorsi dell'istruzione secondaria superiore restano aperti. Resta aperta, ad esempio, la discussione nel Paese e nella politica - l'Unione ha delineato il suo programma al riguardo - su come debba essere la scuola italiana, su quale debba essere il suo ruolo nella vita della società: un'idea della scuola che è tutt'uno con l'idea che abbiamo del Paese, di tutto il Paese, dal Sud al Nord. Già con questo provvedimento, comunque, il Parlamento può comunicare al Paese la volontà di segnare questa fase con i caratteri della serietà, dell'equilibrio, della tensione educativa e culturale. Può farlo con una volontà comune, peraltro già manifestata in Commissione. Continuiamo in molti a pensare che la scuola appartiene a tutti e non certo ad uno schieramento. Vogliamo trasmettere agli studenti un messaggio chiaro: abbiamo fiducia in voi, abbiate fiducia in voi stessi. Siate protagonisti. E allo stesso modo parliamo agli insegnanti: vogliamo sia data dignità alla scuola e al suo lavoro. Attraverso l'esame di Stato il Paese si guarda allo specchio vedendo il suo volto giovane, sognando il suo futuro. Anche attraverso l'esame di Stato il Parlamento sostiene il futuro delle nuove generazioni e anche attraverso l'esame di Stato il Parlamento può mettere in moto l'Italia.

vorrei ricordare la legge n. 62 del 10 marzo 2000, la cosiddetta legge per la parità scolastica.

che sicuramente mi sta ascoltando, sistema nazionale della pubblica istruzione).

Uno dei requisiti per il riconoscimento della parità è che il personale sia fornito del titolo di abilitazione e che i contratti individuali di lavoro rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. giustamente, a mio avviso, ma credo anche ad avviso della stessa relatrice che lo ha puntualizzato, che i docenti delle scuole paritarie devono avere gli stessi requisiti giuridici dei docenti delle scuole statali. legge in esame prevede che i commissari esterni agli esami di Stato siano solo docenti di istituti statali, escludendo completamente da tale possibilità i docenti delle scuole paritarie. Questo è il motivo per cui si pone la questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato,

in quanto, come ho ricordato, fanno parte entrambe del sistema nazionale della pubblica istruzione. Vorrei ricordare, signor Presidente, il dibattito svoltosi del 1999, riportando le parole dell'allora senatore Giaretta - già senatore della Repubblica, da poco dimissionario - che ad un certo punto del suo intervento si lamentava dicendo: «Per la scuola dell'obbligo e per la scuola superiore avremmo preferito un altro strumento, ad esempio quello del finanziamento della funzione docente perché ci sembrava che esso meglio potesse premiare la qualità della scuola, che è quello che ci deve soprattutto interessare». Il senatore Giaretta andava ben oltre la parità prevista dalla legge a suo tempo, come avviene in molti Stati europei, ma ci siamo dimenticati di questo. Non vorrei allora che il comma 4 *sub* articolo 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sia sia stato dettato da quella sinistra massimalista che ha fatto riemergere anche in Commissione vecchi e astiosi rigurgiti di rigido e bieco laicismo nei confronti delle scuole paritarie che, respingendo la legge di parità, le vede ancora relegate a scuole private, soprattutto confessionali, da chiudere specialmente se cattoliche: è questo il motivo per cui vogliamo l'applicazione dell'articolo 93 del Regolamento

una norma debba necessariamente indicare i mezzi per la copertura finanziaria laddove introduca maggiori spese. Un emendamento approvato in Commissione, l'emendamento 1.501, affronta il tema della composizione delle commissioni della maturità prevedendo un'integrazione rispetto alla proposta governativa che con riferimento ai componenti esterni

un'obiezione assai puntuale e stringente. Si era detto sostanzialmente che si faceva un passo indietro, un peggioramento addirittura rispetto alla cosiddetta riforma Berlinguer sulla maturità maturità introducendo un meccanismo che nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto comportare una sorta di scambio di favori e di condizionamento ambientale nella peggiore avrebbe potuto addirittura comportare una discriminazione ai danni della scuola concorrente., trattandosi di commissari che afferivano ad un medesimo bacino di utenza. La relatrice, accogliendo queste nostre osservazioni, ha proposto un emendamento che prevede che i commissari esterni debbano provenire da altri distretti scolastici. Questo emendamento è stato oggetto di un serrato dibattito in Commissione bilancio. Sono state sollevate numerose obiezioni da parte del senatore Enriques, che lo aveva illustrato,

l'emendamento "potrebbe" non determinare oneri superiori. Di fronte poi alle puntuali contestazioni del senatore Vegas, con riferimento in particolare all'esito concernente i Comuni di montagna o Comuni situati in determinate isole, ha ribadito che in tali Comuni non sono "in genere" presentiscuole superiori.

che non vi siano da un distretto all'altro più di 60 minuti, presupposto che renderebbe necessario retribuire ulteriormente i commissari. Ma, al di là di queste considerazioni, c'è da sottolineare che l'emendamento è stato bocciato e respinto dalla Commissione l'emendamento è stato bocciato e respinto dalla Commissione bilancio, a cui si era rimesso il Governo per una valutazione circa la copertura finanziaria. Credo che la Commissione bilancio lo abbia bocciato evidentemente perché non ha avuto alcuna contezza di questa copertura;

la legge potesse essere bocciata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Credo che noi non dobbiamo perdere il nostro tempo e rischiare di approvare una legge che non ha una copertura finanziaria. Dunque, in relazione a quanto definito dalla Commissione bilancio, a cui - ribadisco - lo stesso Governo si era affidato, credo che sia palesemente esistente il problema costituito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Questa legge rischia di non avere copertura finanziaria e dunque non può essere, ai sensi della nostra Costituzione, approvata, ma deve essere rinviata per ulteriori approfondimenti.

alcune considerazioni sulle questioni pregiudiziali che sono state presentate. Vorrei far presente alcuni elementi che ritengo importanti. importanti. L'esame di Stato che andiamo a normare con questo disegno di legge fa riferimento esplicito all'adempimento di un obbligo costituzionale. Proprio per questo, dobbiamo approcciarci

abbiano tali requisiti), avesse contratti di categoria sulla base delle norme di diritto privato, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che normativi. Avevo pensato di poterli inserire quando ho elaborato il disegno di legge, ma - come sapete meglio di me - le scuole paritarie hanno scelto di poter giustamente, nell'ambito della libertà di educazione nel nostro Paese, scegliere i propri docenti sulla base del rapporto fiduciario con dei requisiti condivisi, ma non di accedere al rispetto della Costituzione, che prevede, all'articolo 97, che alle pubbliche amministrazioni si accede per concorso. È questo che impedisce di farlo. Ed è lo stesso motivo cui, anche quando è stata prevista la commissione interna con il solo presidente esterno, in quest'Aula nessuno ha mai sollevato una pregiudiziale motivata dal fatto che il presidente fosse esterno, come non l'avete sollevata neanche questa mattina, perché il combinato disposto tra l'articolo della Costituzione

che dovremmo porre a noi stessi è che non si ripeta mai più - come accaduto in passato, come è successo con il precedente Governo - che gli esami di Stato vengano espletati e ci si dimentichi di pagare i docenti. ritenuto infatti opzionale pagarli, sia in tutto che in parte, affidando alle scuole la decisione se pagare il personale per gli esami di maturità o comprare la carta igienica o quella per le fotocopie.

di spesa, così come previsto, sarà rispettato. Queste sono le motivazioni che ci inducono a ritenere perfettamente legittimo ciò che abbiamo fatto e che abbiamo improntato anche al criterio di serietà, che noi dobbiamo offrire. Ai nostri ragazzi deve essere offerta l'opportunità di avere docenti che dimostrino che l'esame di Stato è un esame serio, meritevole di attenzione e di responsabilità anche nella composizione della commissione, senza porre limiti

sulla questione pregiudiziale presentata dai senatori Asciutti e Davico vorrei, se mi è consentito, spendere qualche parola ulteriore. Il Ministro ha ricordato la norma della Costituzione per cui sarebbe illegittima la partecipazione ad una commissione di concorso da parte di commissari di scuole paritarie perché, il Ministro, ad organismi statali e alla pubblica amministrazione più in generale si accede per concorso. Ma questo non c'entra proprio nulla; e tanto non c'entra che delle commissioni di maturità fanno parte già oggi, già nella proposta del Governo, gli insegnanti delle scuole paritarie come membri interni e non vi è alcuna distinzione tra commissari interni e commissari esterni ai fini della legittima e giuridicamente corretta costituzione della commissione giudicatrice. Se mi è consentito vorrei provare a ribadire alcune delle osservazioni fatte, proponendo anche qualche aggiunta ulteriore. Si diceva correttamente, citando l'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuola statale e dalle scuole paritarie. Dunque, fanno parte del sistema nazionale tanto le scuole statali quanto quelle paritarie. Mi ricorda l'articolo 1 una famosa definizione presente nelle fonti romane che sicuramente il senatore Brutti ben conosce: "*Iura popoli romani constant ex*". *definitio* *per partes*; il tutto, l'insieme: il sistema nazionale della scuola; le sue parti, le parti che compongono il tutto: la scuola statale e la scuola paritaria.

che non abbiano chiesto la parità sono escluse; stanno al di fuori; sono - come si direbbe, ricorrendo ancora a terminologia romanistica - *extra ordinem*. La parità indica un rapporto di equivalenza; sono pari; sono in un rapporto di equivalenza. E non a caso tutti, a prescindere dall'orientamento, possono accedere a questa scuole: ogni giovane, ogni ragazzo può iscriversi senza preclusione di sorta. D'altro canto, se abbiamo sottolineato come vi sia una totale parità, come entrambi questi modelli di scuola facciano parte di un unico sistema, i docenti anche nelle scuole paritarie devono essere abilitati; devono avere un'abitazione nazionale. Sono dunque posti nelle stesse condizioni giuridiche dei docenti delle scuole statali. E questo perché? Sia le scuole paritarie private sia le scuole statali, come specifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, svolgono un servizio pubblico. È abbastanza singolare un altro fatto, che i docenti delle scuole paritarie possono far parte delle Commissioni di maturità, come commissari interni. Possono dunque legittimamente costituire una commissione d'esame possono contribuire a rilasciare un titolo, avente valore legale: lo Stato, l'ordinamento nazionale conferisce a questi docenti il potere di contribuire a conferire un titolo avente valore legale. Questi docenti hanno un identico titolo giuridico. Se a questo punto dovessero essere esclusi, ipotesi perché hanno una caratterizzazione religiosa, dalla possibilità di far parte anche delle commissioni come commissari esterni, si violerebbe certamente la nostra Costituzione che prevede che non ci possano essere discriminazioni in ordine all'appartenenza, alla fede, alla confessione religiosa che viene professata. Allora perché dovrebbero essere discriminati? Perché dovremmo trattare come docenti di serie B questi insegnanti insegnanti abilitati, che insegnano in scuole che fanno parte di un unico sistema, poste su un piano di parità, che già possono far parte legalmente, possono costituire giuridicamente le commissioni di concorso per gli esami di maturità? Credo dunque che sia palesemente incostituzionale una norma di questo tipo, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Ma vi è poi anche una contraddizione nello stesso provvedimento del Governo perché, se è vero che esclude questi soggetti dalla composizione delle commissioni, tuttavia vi è un ordine del giorno approvato in Commissione che impegna il Governo e da questo è stato accettato, a promuovere iniziative di formazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, ma anche dei docenti e dei dirigenti delle scuole paritarie ai fini appunto dello svolgimento delle funzioni di commissario d'esame per la maturità.

delle commissioni giudicatrici; dopo di che si contraddice. Ecco allora perché chiedo - e sono d'accordo - che sia bocciato ai fini della costituzionalità il provvedimento.

credo che l'opposizione abbia dato dimostrazione di grande senso di responsabilità: alla Camera si sta discutendo una pessima finanziaria che opera il più grande taglio di risorse mai fatto sulla scuola italiana, smentendo tutte le promesse dell'Unione in campagna elettorale;

con un aumento dell'obbligo scolastico, senza peraltro stanziare risorse adeguate per poterlo attuare. Il ministro Fioroni, di fronte alle nostre puntuali contestazioni, convincenti in Commissione, dimostrando di non avere ben chiare le cifre e l'impatto della finanziaria sulla scuola italiana. In un quadro di questo tipo, avremmo potuto disinteressarci del provvedimento oggi in discussione, lasciando che la maggioranza si arrangiasse

diversamente da quanto ha fatto il centro-sinistra nella passata legislatura. Abbiamo cercato dunque di migliorare, laddove possibile, il progetto - senz'altro inadeguato e carente - presentato dal Governo. La maggioranza ha accolto alcuni nostri emendamenti, alcuni di contorno ed altri di sostanza. Diamo atto alla relatrice di avere trattato con equilibrio ed attenzione il rapporto con l'opposizione, pur costretta nella camicia di Nesso confezionatale dal suo Governo e dalla sua composita maggioranza. Proprio le profonde divisioni manifestatesi all'interno della coalizione di Governo, emerse con chiarezza nel dibattito in Commissione, hanno impedito che, al di là di qualche miglioramento su singoli punti dovuto essenzialmente al contributo dell'opposizione, si potesse migliorare in modo significativo l'intero disegno governativo. Dunque, viene portata in Aula una maturità nel suo complesso incolore, sostanzialmente modesta, che ritorna nello spirito alla riforma Berlinguer del 1998, pur recependo qualche novità, peraltro già contenuta nel decreto Moratti sulle superiori o ispirata - appunto - dagli emendamenti dell'opposizione. Così lo scrutinio di ammissione era stato abolito dal centro-sinistra nella XIII legislatura ed era stato invece reintrodotto già nel decreto Moratti sul II ciclo. Ilpotenziamento del rapporto con l'università sta già nella legge 28 marzo 2003, n. 53, e nel decreto attuativo ed ha lì un'ampiezza ed un'organicità ben maggiori. La necessità di recuperare tutti i debiti pregressi è contenuta nella citata legge n. 53, tanto da prevedersi che, se al termine del quarto anno non si siano saldati i debiti, non si sarà ammessi all'anno successivo. La norma sugli "ottisti", che vuole scoraggiare i diplomifici, era già contenuta sempre in quel decreto Moratti che voi avete sospeso. La proposta del ministro Fioroni era semmai piuttosto indulgente: accogliendo un emendamento di Alleanza Nazionale e di Forza Italia si sono resi un po' più severi i criteri di valutazione; forse potevate avere più coraggio, come vi chiedeva un emendamento specifico di AN. La vera novità che caratterizza questa riforma rispetto al decreto Moratti sul secondo ciclo è il ritorno dei commissari per metà esterni: la soluzione che avete accolto appare tuttavia ispirata dalla logica del "vorrei, ma non posso". Avete dato vita a qualcosa di stiracchiato, di inadeguato, di provvisorio, lo si intuisce persino tra le righe di alcuni vostri interventi. Avete comunque rieditato una formula che ha già dimostrato in passato di non funzionare. È proprio questo è il punto: rispetto alla maturità Moratti, con tutti i membri interni, la maturità Berlinguer, con la metà dei commissari esterni, non determinò esiti diversi. Basta considerare le cifre: cento di promossi nel 2001 e addirittura qualcuno in meno nel primo anno di applicazione della Moratti (95,7 per cento), che vide poi attestarsi i promossi sul 96,5 per cento negli anni successivi. Ma allora occorre essere chiari: l'inserimento dei commissari esterni si giustifica solo perché dovrebbe consentire una valutazione più oggettiva, possibilmente meno indulgente; la sostanziale identità degli esiti induce a porre una prima domanda non trascurabile: vale la pena spendere quasi 150 milioni di euro quando i risultati sono gli stessi? però, non sono nemmeno questi i risultati che vi interessano, se è vero come è vero che in finanziaria avete incoraggiato i docenti italiani a diminuire le bocciature del 10 per cento per risparmiare 130 milioni di euro in tre anni. anni. Ma se non si ha il coraggio di cambiare in modo significativo questa maturità, non sarebbe meglio allora destinare questi 150 milioni di euro, o quasi, alla riduzione dei tagli sulla scuola contenuti nella finanziaria, alla valorizzazione dei docenti, alle spese di autoaggiornamento degli stessi o alla stessa edilizia scolastica, i cui fondi non sono mai abbastanza? Si vari piuttosto la riforma Moratti del secondo ciclo, che conteneva già la gran parte delle poche cose positive contenute in questo disegno di legge. Alleanza Nazionale fin dall'inizio del dibattito aveva posto tre condizioni per dare il proprio assenso ad una riforma della maturità: una terza prova organizzata e gestita da un ente esterno; i commissari tutti esterni, tranne il membro di garanzia; la verifica del possesso delle basi culturali generali riferite all'intero percorso scolastico e non solo un accertamento delle competenze riferite all'ultimo anno. Avevamo anche espresso riserve su punti più specifici, come, per esempio, la possibilità per gli studenti extracomunitari che non abbiano frequentato l'ultimo anno di essere ammessi direttamente all'esame di maturità con un regime agevolato rispetto agli studenti italiani, così come era invece previsto nel testo originario del disegno di legge. Più in generale abbiamo chiesto un cambiamento di indirizzo e di visione culturale: chiedevamo una riforma della maturità che fosse occasione per ridare serietà all'intero percorso scolastico, che ripristinasse l'idea di una scuola come luogo dove si studi seriamente, in cui si privilegi chi nel percorso scolastico ha assunto un atteggiamento di responsabilità e di impegno; ma per far ciò si devono, in primo luogo, dare gli strumenti per una verifica oggettiva, il più possibile terza, al termine del percorso. *(Brusìo)*. Chiederei però un po' di silenzio, anche dai senatori

Siamo l'unico Paese al mondo dove la promozione appare un diritto, dove si ha timore ad usare il termine "selezione", dove sono ancora consentite le occupazioni delle scuole. Come è allora possibile non tener conto del fatto che, per esempio, alcune settimane siano state da taluni sprecate nella perpetuazione di stanchi riti che costituiscono pur sempre reati? Credo sia ora di dire basta ad un modello di scuola facile, indulgente, non formativa anche nel carattere, incapace di premiare il merito; abbiamo bisogno di una scuola che aiuti a formare persone adulte, non eterni adolescenti. Quando faccio i confronti con quello che accade all'estero c'è da preoccuparsi. In questo contesto occorre poi la consapevolezza che il compito della scuola finisce con lo scrutinio di ammissione, la maturità è la verifica che fa lo Stato della preparazione complessiva dello studente per potergli attribuire un titolo avente valore legale. È lo Stato che attribuisce il valore legale ad un titolo, non la scuola. Ecco perché è fondamentale che la terza prova sia gestita esternamente: si sarebbe trattato di un momento di valutazione oggettiva, senza possibilità di fare sconti, una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Ecco inoltre perché abbiamo chiesto che i commissari fossero tutti esterni e non venissero dallo stesso territorio dei membri interni. Ecco perché abbiamo tanto insistito sulla verifica delle basi culturali generali. Delle nostre tre condizioni solo una è stata accolta. Quanto meno ora, grazie ad un emendamento di Alleanza Nazionale, si definisce a cosa serve l'esame di maturità: nel testo del Governo non era nemmeno specificato. Grazie al nostro emendamento si concepisce dunque il percorso formativo come un tutto unitario, in cui l'ultimo anno appare come il completamento di un intero percorso, non come qualcosa di isolato. Abbiamo anche apprezzato l'emendamento della senatrice Capelli che in qualche modo è venuto incontro alle ragioni della nostra contrarietà al testo originario del Governo che determinava una oggettiva disparità di trattamento fra studenti italiani ed extracomunitari, garantendo a questi ultimi inammissibili scorciatoie. Non vi è stata tuttavia quella svolta che chiedevamo: sulla terza prova sono emerse tutte le contraddizioni della maggioranza. Al riguardo, il senatore Ranieri ha dichiarato che si tratterebbe di «un compromesso che cerca di tenere insieme Capelli e Valditara», ma si tratta ma si tratta di un compromesso pasticciato. Cito qui proprio la senatrice Capelli che parla di «risultato confuso, inadatto a svolgere» i compiti che si vorrebbe prefiggere. Insomma per una parte della maggioranza sarebbe un modo inadeguato, pasticciato di «venire incontro alle sollecitazioni dell'opposizione», con riferimento al discorso della terza D'altro canto era noto che la terza prova sarebbe stata la cartina di tornasole della vostra reale volontà riformista. So che alcuni di voi non hanno posizioni molto distanti dalle nostre, su questo punto. Avete tuttavia dovuto subire il condizionamento della CGIL e di una parte della maggioranza che sull'emendamento che avete proposto che avete proposto lamenta addirittura la lesione della autonomia scolastica e delle prerogative del Parlamento. In realtà avete al vostro interno componenti allergiche a qualsiasi idea di verifica dei risultati e di valutazione esterna, difensori strenui di un concetto autoreferenziale, non meritocratico, sostanzialmente irresponsabile di scuola. Un risultato comunque l'abbiamo ottenuto: fino ad agosto sembrava che l'INVALSI dovesse sparire, che la valutazione esterna fosse un tabù, ora ridate un ruolo all'INVALSI e, pur fra mille cautele, lasciate intravedere l'idea di una valutazione dei risultati. Peccato che ancora una volta abbiate scelto la logica del «vorrei, ma non posso». Vi è mancato il coraggio, avete sprecato una importante occasione in nome della unità della vostra coalizione. Come non comprendere infatti che il ruolo che affidate a questo INVALSI non è molto diverso da quello di un qualsiasi istituto che predispone modelli: in definitiva si pone sullo stesso piano dell'IPSOA! La scuola se ne può bellamente infischiare dei modelli prodotti dall'INVALSI e, soprattutto, non vi è alcuna garanzia di una oggettività e di una omogeneità di questa terza prova per tutte le scuole, su tutto il territorio nazionale. Avete scelto di privilegiare la forma, sulla sostanza. A che serve una prova gestita tutta internamente alla scuola? La scuola ha avuto cinque anni per valutare il ragazzo, e il suo giudizio lo ha dato al momento dello scrutinio. Veniamo ai commissari esterni: voi avete riconosciuto che una commissione composta tutta da esterni sarebbe stata la soluzione migliore, e avete anche riconosciuto che i commissari esterni non possono provenire dal medesimo Comune. Al riguardo vi do atto di aver compiuto un gesto di onestà intellettuale accogliendo un mio ordine del giorno, firmato anche dal senatore Ranieri, in cui si invita il Governo a reperire risorse per far sì che i commissari esterni provengano almeno dall'ambito regionale, riconoscendo implicitamente l'inadeguatezza della soluzione proposta dal Governo. Avete obiettato tuttavia che non vi sono le risorse per fare meglio: ma allora è lo stesso ragionamento che spinse nella scorsa legislatura verso quella commissione tutta interna che voi avete così tanto esecrato e che, come si è visto, ha dato risultati sostanzialmente analoghi alla riforma che voi proponete. ritorna ancora una volta la logica del «vorrei, ma non posso». Per venire incontro alle nostre critiche avete stabilito che i commissari esterni non devono provenire dallo stesso distretto: ma questo è il ritorno alla riforma Berlinguer, nel testo del Governo vi era una soluzione persino peggiore della Berlinguer, addirittura un grave passo indietro. Come non rendersi conto infatti che reclutare i commissari esterni nello stesso Comune in cui si trova la scuola avrebbe creato più danni che benefici: nella migliore delle ipotesi avrebbe favorito una logica di scambio; nella peggiore si sarebbe corso il rischio di rivalse per danneggiare la scuola concorrente. E tuttavia anche questo minimo, scontato miglioramento è a rischio: l'emendamento della relatrice è stato bocciato dalla Commissione bilancio perché non sarebbe sicura la copertura finanziaria. E questo è un passaggio grave. Vi è anzi da chiedersi se dopo i pesanti tagli alla scuola che prevedete in finanziaria vi saranno ancora risorse per reperire quei quasi 150 milioni di euro necessari per pagare i commissari di concorso oppure farete come state facendo per l'obbligo scolastico: riforme senza soldi. Ma vi è un ulteriore passaggio che ci ha lasciato perplessi e proprio nell'intervento conclusivo del Governo in Commissione. La vice ministro Bastico, riconoscendo la bontà di alcune nostre proposte, in particolare in relazione alla struttura della terza prova, ha testualmente dichiarato che potranno essere meglio considerate quando si farà la riforma delle superiori, rinviando dunque ad una riflessione ulteriore da farsi in quella occasione. Ha così concluso che in questo disegno di legge vi sarebbero solo aggiustamenti in attesa di una riflessione ulteriore da compiersi in occasione della preannunciata riforma del secondo ciclo, sottolineando peraltro come ciò che noi proponiamo si collocherebbe su una medesima linea di tendenza. Ma allora che razza di riforma è mai questa che stiamo discutendo oggi? Mi pare dunque di capire che rischiamo di dare vita all'ennesima riforma provvisoria della scuola italiana, a qualcosa che già si preannuncia dovrà essere ripensato e probabilmente migliorato. Si tratterebbe dunque di una riforma transitoria che già si ipotizza di cambiare. Ma la scuola italiana, gli studenti italiani sono stanchi di riforme provvisorie. Più organicamente, il precedente Governo aveva previsto di cambiare la maturità insieme con la riforma delle superiori, in quel decreto che voi avete invece sospeso. È evidente, a questo punto, che questa riforma risulta come sospesa per aria, senza solide basi. Vi è poi un altro punto, l'ennesimo, su cui sono affiorate le vostre contraddizioni e alla fine ha prevalso, come sempre, uno spirito conservatore, statalista e poco liberale. È stupefacente la vostra posizione sulle paritarie: proponente un ordine del giorno in cui s'invita lo Stato a formare anche i docenti delle scuole paritarie insieme con quelli delle scuole statali, in vista della partecipazione alle commissioni di esame in veste di membri interni e poi non riconoscete a questi docenti anche il ruolo di commissari esterni, dunque li considerate inadeguati, all'interno del sistema pubblico di istruzione create una categoria di docenti di serie B; francamente, mi interessano poco le vostre giustificazioni, avete detto: «non possiamo spaccarci ». Insomma, per l'ennesima volta, rivelate di essere come Giano bifronte: un viso che guarda avanti e l'altro che guarda all'indietro e ancora una volta è quello che guarda indietro che alla fine ha avuto la meglio. Nonostante qualche miglioramento, questa riforma non risponde, dunque, ad un'idea moderna di scuola e temo che non contribuirà a risolvere quella che appare una delle maggiori critiche che si leggono nelle periodiche relazioni dell'OCSE: la eccessiva facilità e la sostanziale deresponsabilizzazione del nostro modello di istruzione. Con i vostri innumerevoli «vorrei ma non posso », voi dimostrate che ciò che manca non è la consapevolezza dei problemi, ma la inadeguatezza del vostro Governo, che non ha volontà e spirito per trasformare le parole in fatti concreti.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi senatori, intervengo a favore del provvedimento in esame ed auspico che, come già avvenuto nel corso del confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo, anche in quest'Aula si realizzi il più ampio consenso sul provvedimento che contiene le disposizioni in materia di esami di Stato. L'istituzione scolastica ha rappresentato un cardine essenziale nella crescita del nostro Paese, un punto di riferimento irrinunciabile per intere generazioni di donne e di uomini che hanno costruito il tessuto produttivo, intellettuale e materiale italiano. È questo il ruolo che abbiamo il dovere di riguadagnare all'istituzione scolastica. Un ruolo che è culturale e, nello stesso tempo, sociale. Il processo di svalutazione dell'istruzione cui abbiamo assistito in questi ultimi anni - al quale hanno concorso, seppure inintenzionalmente, il sistema mediatico, la famiglia, la scuola e la politica stessa si traduce nell'enfasi posta sul successo, piuttosto che sull'impegno, sul possedere e sull'apparire piuttosto che sull'essere, sull'informazione piuttosto che sulla formazione. All'interno delle famiglie si rileva una quasi totale sfiducia nella competenza delle istituzioni scolastiche a supportare processi decisionali e si preferisce, per prendere decisioni importanti per il futuro, sia formativo che lavorativo, muoversi esclusivamente all'interno di reti circoscritte e tradizionali (le parentele e le relazioni amicali). Tutto ciò segnala una profonda distanza, oltre che un profondo senso di sfiducia, nei confronti delle istituzioni. La sfiducia delle famiglie si riversa fatalmente sui giovani, alimentando un deleterio circolo vizioso che delegittima l'istituzione scolastica, privandola di quel riconoscimento di competenza essenziale per portare a termine con efficacia il compito educativo. È veramente molto significativo che il primo provvedimento proposto dal Governo alla discussione parlamentare sia centrato sull'obiettivo di restituire nuova credibilità e autorevolezza agli esami di Stato. Si tratta di un momento dal forte valore simbolico: rappresenta la chiusura di un percorso di studi, ma anche un formativo rituale di passaggio, che segna il percorso verso l'età matura della consapevolezza e della responsabilità individuale. Riguadagnare attraverso questo provvedimento la serietà e l'importanza di tale momento significa contrastare il rischio della perdita di valore legale del titolo di studio e le sue conseguenze in un mercato del lavoro sempre più esigente. Significa restituire valore al lavoro scolastico dei nostri giovani e dei loro insegnanti, anche attraverso il contrasto dei cosiddetti diplomifici, specializzati nel far ottenere esiti brillanti - se così possiamo dire - a privatisti senza merito. Ma significa anche segnare la volontà di un'inversione di tendenza nelle dinamiche sociali e nei valori condivisi dalla comunità, tale da permettere di recuperare di recuperare il senso dell'esito finale come reale riconoscimento del percorso di istruzione svolto e dell'impegno profuso. Significa dare al nostro Paese un primo strumento reale per colmare il divario - in qualità, equità e meritocrazia - che separa la nostra scuola da quelle delle Nazioni industrializzate al nostro pari. Ma è sul concetto di equità che vorrei richiamare la vostra attenzione, in ragione delle prospettive che il provvedimento oggi in esame delinea per il futuro della scuola italiana. È indubbio che sia necessario - direi vitale per l'istituzione scolastica - attuare politiche di rafforzamento della qualità e della serietà dei percorsi formativi, favorendo la responsabilità degli studenti e di tutti gli operatori scolastici. Parimenti, non possiamo ignorare quanto il contesto sociale di provenienza assuma, ancora oggi, un peso preponderante nel determinare il successo scolastico: gli studenti con un più basso livello socio‑economico risultano avere prestazioni tre volte più povere rispetto agli appartenenti a classi sociali più elevate. Ancora oggi si rileva una variabilità troppo altra tra differenti scuole, anche nella stessa area geografica, per quanto riguarda la qualità e l'efficacia dei processi formativi. Ciò condiziona pesantemente le opportunità dei giovani e, di conseguenza, lo sviluppo dell'intero nostro sistema produttivo. Ciò depotenzia il ruolo e l'immagine della scuola, troppo spesso percepita come un limite piuttosto che come un'opportunità. La Campania e il Mezzogiorno, territori pesantemente segnati da antiche e nuove criticità, vivono in modo drammatico queste diseguaglianze. Nell'anno scolastico 2005-2006, il tasso di dispersione in città quali Napoli e Palermo ha oltrepassato il 40 per cento (contro una media nazionale, già fin troppo alta, del 32 A Napoli soltanto una scuola su cento realizza il prolungamento di orario, il cosiddetto tempo pieno: a Milano l'88 per cento! Sono dati impressionanti che definiscono i contorni di un profondo divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese. Trovo importante e significativo che le alte cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica, abbiano sentito la necessità di ribadire con forza l'unità del Paese quale valore costituzionale fondante della nostra democrazia. Nondimeno, bisogna prendere atto di come - nei fatti, nella realtà del Paese, nella vita quotidiana dei cittadini - l'accentuazione sempre più marcata del divario Nord-Sud rischi di determinare i contorni di un vero e proprio processo di secessione nascosta e strisciante. I giovani meridionali patiscono forti diseguaglianze di opportunità, proprio nel momento più delicato della propria biografia di formazione. Ancora in queste ultime settimane, così drammatiche per la città di Napoli, in più occasioni il Governo ha dichiarato l'impegno a favorire l'apertura pomeridiana delle scuole quale fattore concorrente a una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata e al tessuto economico parallelo e illegale che rappresenta un male storico della città, con esiti e ricadute devastanti sul tessuto sociale. La reale efficacia di tale proposta, già sostenuta con i mezzi e le risorse delle istituzioni locali, si misurerà sulla volontà e la capacità di costruire processi concreti e reali di impegno e coinvolgimento di studenti, insegnanti, famiglie e forze attive sul territorio. È necessario un investimento forte e costante per restituire qualità all'istituzione scolastica, autorevolezza agli insegnanti e capacità di interessare i giovani con attività realmente coinvolgenti. Se non sarà supportata da strumenti e risorse adeguate, l'apertura pomeridiana e serale delle scuole napoletane rischia di rimanere uno *slogan*, efficace ma privo di reale forza di cambiamento, potrebbe addirittura generare un doposcuola di serie B, di cui la città non sente il bisogno, avendo inoltre chiare le conseguenze ancora più devastanti che un intervento limitato, semmai frettoloso, può avere in una situazione così complessa e drammatica. Bisogna investire, molto e molto di più, per la scuola napoletana e meridionale e per farlo è necessario conoscere, rispettare, valorizzare ed estendere le esperienze che hanno già dato tanti buoni risultati, costruendo insieme con il territorio e gli operatori quel percorso virtuoso che potrà dare i frutti sperati. Proprio in ragione di una situazione fortemente compromessa, negli ultimi anni Napoli e la sua Provincia sono stati teatro di una profonda riflessione su questi temi, che ha già portato alla realizzazione di tante esperienze positive, che delineano concretamente quella scuola cosiddetta della seconda opportunità, necessaria per fronteggiare situazioni particolarmente critiche, ma utile anche per l'attuazione di più efficaci pratiche di integrazione. Desidero richiamare brevemente almeno tre esperienze. La prima è il progetto «Chance», definito e conosciuto come quello dei «maestri di strada», che da molti anni riesce a contrastare la dispersione scolastica e a recuperare alla scuola (strappandoli alle attività criminose) decine di ragazzi che hanno ripreso dignità, ottenuto la licenza media, fatto sport e musica. Si è riusciti a rendere attraente la formazione, a non far percepire la scuola come un nemico; i ragazzi hanno partecipato anche a esperienze di lavoro protetto, ma non simulato. tutti i progetti di tutoraggio da parte dei ragazzi più grandi della stessa scuola, finalizzati a stabilire ponti culturali più larghi verso gli alunni, coinvolgendoli in tante decine di attività e anche coinvolgendo le loro madri, le scuole aperte il pomeriggio alle mamme nei quartieri più degradati e poveri, quelle mamme che non hanno nessuna opportunità e che diventano appunto elemento di tutela del processo formativo per i loro ragazzi. Vorrei ricordare inoltre le tante esperienze di educazione alla legalità: penso all'istituto superiore «Rosario Livatino», nella periferia orientale, la prima scuola italiana dove la cultura della legalità è divenuta materia d'insegnamento, al pari della matematica o dell'italiano, e non è attività accessoria. Ogni giorno, 1.200 ragazzi dedicano una quota delle loro ore di studio all'approfondimento della Costituzione, all'esame critico dei giornali, alla discussione sui principali fatti di cronaca. In generale, quello che emerge dall'esperienza napoletana è la possibilità concreta di costruire una nuova personalità e un nuovo statuto deontologico degli studenti e delle studentesse. È necessario però che le esperienze positive escano dagli ambiti della precarietà e dell'eccezionalità: devono diventare pratica istituzionale condivisa, *modus* *operandi* integrato nelle politiche formative nel loro complesso, patrimonio comune che assume dignità ai fini della valutazione conclusiva. In questa direzione spinge il provvedimento oggi all'esame di questa Assemblea. Il nuovo esame di Stato, ripristinando il giudizio di ammissione da parte del consiglio di classe, restituisce a ogni singola scuola la responsabilità, la dignità, l'autonomia per valorizzare, anche attraverso l'istituto dei crediti formativi, il lavoro svolto in ragione del superamento di condizioni di svantaggio e l'impegno nella costruzione di coscienza civile e sociale. È necessario spingere la scuola a riappropriarsi del suo ruolo di «costruttore» dell'identità civile del nostro Paese e di punto di riferimento, non soltanto per i giovani, ma anche, e sempre di più, per le loro famiglie. La scuola italiana, con la sua competenza, deve avere tutti gli strumenti necessari ad accompagnare il Paese verso un maggiore e più armonico sviluppo. Una scuola fondata sui diritti inalienabili dell'individuo, sui criteri di qualità ed equità, sarà la scuola democratica e competente di cui il nostro Paese ha bisogno per crescere. Diceva Giovanni Falcone: «Solo un esercito di maestri potrà sconfiggere un giorno la criminalità». Io penso che quel giorno è arrivato, penso che possiamo provarci, però dobbiamo crederci tutti. Tutti e tutte e, credo, anche quest'Aula - maggioranza e opposizione - possiamo avere fiducia nelle parole e nel testamento morale di Giovanni Falcone.

il disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea nasce dall'esigenza di contemperare diversità di accenti e di convinzioni, di princìpi e di mentalità, di opinioni e di vedute fra le varie forze politiche in ordine ai processi che governano la scuola di oggi. Il problema della struttura e della funzione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria, si è imposto ormai da tempo con il maturare della consapevolezza che non è più possibile ignorare l'evoluzione delle esigenze che ha accompagnato lo sviluppo storico della nostra società. In questo senso l'esame di Stato - non vi è dubbio - si configura come uno tra i temi più delicati dibattuti all'interno del comparto della pubblica istruzione; per il fatto che esso costituisce il momento di centralità formativa dell'intero nostro sistema scolastico. Certo, l'atteggiamento di ostilità e di rifiuto da parte del ministro Fioroni e del suo *staff* di Vice Ministri e Sottosegretari nei confronti di ciò che di moderno e innovativo è stato introdotto dal precedente Esecutivo nella scuola, non depone positivamente ai fini di un sereno ed equilibrato confronto democratico tra maggioranza ed opposizione. L'atteggiamento del Ministro e i suoi giudizi di merito sui processi che hanno caratterizzato la scuola negli ultimi cinque anni fanno perno e si sostanziano di una filosofia e di un programma di Governo, a dir poco, minimalista, secondo cui in materia di rinnovamento scolastico è meglio abrogare che riformare la precedente normativa. Da qui l'idea ossessiva che finora lo ha contraddistinto: quella cioè di un capillare «smontaggio» della riforma Moratti attraverso dissennate dichiarazioni volte a cancellare i cardini su cui s'incentra la legge 28 marzo 2003, n. 53, e attraverso continue circolari ministeriali dirette a suggerire comportamenti del tutto difformi dalla legislazione vigente. Un tale comportamento, unito a un maldestro tentativo di ripristino della vecchia strutturazione degli esami di Stato, riporterebbe indubbiamente indietro di venti anni le lancette dell'orologio della scuola italiana. Occorre invece maggiore apertura, maggiore flessibilità, maggiore disponibilità al dialogo e al confronto con le parti politiche; cosa che all'interno della 7a Commissione permanente, per fortuna, è possibile riscontrare anche quando le soluzioni non raggiungono l'obiettivo della convergenza e dell'unità. Il dibattito in Commissione, dunque, su questo delicatissimo tema c'è stato. È stata una discussione incalzante, a volte spigolosa, animosa, ma essenzialmente improntata a un corretto e civile confronto democratico. Confronto caratterizzato, ovviamente, da alcuni punti fermi di comune convergenza, quali l'esigenza di maggior rigore e serietà dell'esame; le finalità cui tende la verifica conclusiva nella secondaria superiore; il contesto nel quale si colloca il nostro sistema d'istruzione, che è quello dell'articolo 33 della Costituzione, relativo alla libertà d'insegnamento e al particolare compito dello Stato di poter istituire scuole statali e di dettare le norme generali sulla parità scolastica. E tuttavia, nonostante i tentativi condivisi di miglioramento del disegno di legge in Commissione, esso presenta ancora delle criticità che vanno ora affrontate in Assemblea. Naturalmente puntare a un maggior rigore nella valutazione scolastica è giusto, ma non dimentichiamo che tale obiettivo è stato quello che si è sempre perseguito nelle leggi di riforma della XIV legislatura. Così come, del resto, è giusto, dal punto di vista educativo, attuare un sistema di valutazione rigoroso e graduale, interno ed esterno, capace di verificare i livelli di apprendimento dello studente, soprattutto nei bienni che precedono l'ultimo anno, al fine di consentire il recupero graduale degli insuccessi scolastici all'interno del biennio, pena la non ammissione a quello successivo. In questo senso, sia pure con sensibilità diverse, si è verificata una sostanziale convergenza in Commissione; come pure sulla necessità del ripristino dei requisiti di ammissione incautamente cancellata dalla riforma Berlinguer del 1997 e ridotta semplicemente alla frequenza dell'ultimo anno. Voglio ricordare al riguardo un dato storico: nel 1998, quando non era ancora in vigore la riforma Berlinguer, la percentuale dei non ammessi oscillava tra il 6 e il 7 Ebbene, l'anno successivo il 1999 anno di entrata in vigore della riforma che cancellava dallo scrutinio finale l'ammissione all'esame, i promossi passarono dal 92 al 97 per cento dei candidati, con grande sdegno di Berlinguer. Il che conferma la tesi del grosso abbaglio preso dal Ministro di allora che in nome della trasparenza e serietà dell'esame, si era forse lasciato andare al populismo demagogico del «tutti ammessi, tutti bravi, tutti promossi». Ma tornando al disegno di legge in esame, l'introduzione di nuove norme tese a garantire maggiore trasparenza e maggior rigore per i candidati interni ed esterni ha fatto riemergere vecchi ed astiosi rigurgiti di rigido e bieco laicismo, come ho già detto poc'anzi,

e non dimenticare che la legge sulla parità fu fatta da un analogo Governo di centro-sinistra nei cinque anni che hanno preceduto la precedente E questo non è giusto. A scanso di ogni equivoco, ritengo di poter affermare che tutti - credo - tutti siamo contro i «diplomifici»; perché essi sviliscono la qualità dei processi didattico-educativi, cancellano un serio e normale *iter* scolastico, ostacolano un naturale svolgimento dell'istruzione e formazione della cultura. E tuttavia, con i provvedimenti normativi che il Parlamento si è dato in questi anni - mi riferisco *in primis* alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica - credo sia giunto davvero il momento di rimuovere questo sterile pregiudizio, tipico di una certa sinistra, secondo cui le scuole paritarie rappresenterebbero l'erba selvaggia da estirpare nel giardino fiorito di una scuola tutta statale. Vorrei ricordare al Ministro che l'articolo 97 della Costituzione riguarda

dello Stato italiano, non di ruolo, assolutamente: li possiamo anche elencare, dai Beni culturali alle Università e così via. Ma probabilmente il Ministro non aveva altre risposte e ha fatto riferimento all'articolo 97; forse la Costituzione va utilizzata diversamente. Le scuole paritarie (dobbiamo mettercelo bene in testa), come tutte le altre scuole, sono scuole pubbliche che offrono un servizio - quello scolastico-formativo - a cui tutti possono e devono essere liberi di accedere. Nel ribadire, dunque, la mia ferma contrarietà nei confronti dei «diplomifici», intendo anche precisare che tale deprecabile fenomeno non deve risolversi a danno delle scuole paritarie più serie. Al contrario, è preciso compito del Governo utilizzare gli strumenti offerti dalla legge n. 62 del 2000 per revocare eventualmente la parità agli istituti che abbiano dimostrato di non meritarla. Ma il Governo questo coraggio non ce l'ha: preferisce un provvedimento legislativo come quello in esame, per nascondere la volontà di eliminazione della parità scolastica. Il nostro disegno di legge, in questo senso, prevede sistematiche e costanti verifiche sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari. In coerenza con esso, perciò, riteniamo che la organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, vengano assicurati nell'ambito di un rigorosa operatività della funzione ispettiva. Nel confronto, dunque, che ha caratterizzato la Commissione, al di là del comune accordo di proseguire nel cammino di riforma e modernizzazione del sistema scolastico già avviato, al di là, inoltre, dell'intesa di incentivare il merito degli studenti nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le posizioni tra maggioranza ed opposizione su alcuni punti sono rimaste distanti. Su due nodi fondamentali, in particolare, le nostre analisi non si sono ritrovate con quelle della maggioranza: ovvero sull'alta percentuale di promossi e sulla composizione della commissione esaminatrice; senza dubbio, due essenziali elementi indicatori della progressiva china e perdita di serietà dell'esame di Stato. Relativamente alla prima analisi: da tutti i dati rilevati risulta che dall'avvento della scuola di massa il problema della «serietà» ha poco o nulla a che fare con la composizione delle commissioni. Dopo la riforma del 1969, si sono avute tre tipologie di commissioni: tutta esterna con il solo commissario interno; metà esterna e metà interna; tutta interna con il presidente esterno. I promossi con le tre combinazioni variano dal 95 al 98 per cento. Il problema, allora - come ho avuto modo di spiegare in Commissione - è altrove e occorre individuare i veri nodi della questione. Se per alta percentuale di promossi s'intende l'inequivocabile necessità di tornare a un esame severo, erudito, selettivo, certamente il disegno di legge del Governo non ci trova sulla stessa lunghezza d'onda; visto che, in realtà, la questione centrale - dopo la scolarizzazione di massa che ha interessato il nostro sistema scolastico a partire dagli anni Settanta - non sta più soltanto in un problema di selezione fine a se stessa. Né è pensabile che sia ancora possibile appigliarsi alla questione del valore legale del titolo di studio, dal momento che - pur riconoscendo che i titoli conferiti dagli istituti superiori superiori continuano ad avere valore legale in quanto producono effetti giuridici consentendo la prosecuzione degli studi, la partecipazione a concorsi pubblici e, qualche volta, l'inserimento nel mondo del lavoro - in effetti il vero problema non sta, né va semplicemente rintracciato nel *curriculum* o nella votazione conseguita, ma nella qualità delle conoscenze possedute dagli studenti e nelle esperienze *post*-scolastiche.

non va); il che farebbe pensare a un eccellente livello di preparazione dei giovani. Non è così. O almeno: il nostro convincimento e le nostre conclusioni non sono di questa natura. Le indagini OCSE, signor Presidente, fotografano infatti una realtà ben diversa, a testimonianza di criticità ben più a monte rispetto agli esami di maturità. Cosa intendo dire? Voglio dire che la pur conclamata esigenza di rigore non va rivolta tanto al termine dei corsi di studio, quanto piuttosto a tutto l'arco della loro durata, dedicando particolare attenzione all'effettivo superamento dei debiti formativi. In questo senso ritengo, e ne sono manifestamente convinto, che solo superando un certo lassismo e permissivismo culturale - che oggi, per certi versi, pervade la scuola, con particolare riguardo a tutto il percorso scolastico e non ad un solo anno - si potranno produrre competenze certificabili e spendibili per una efficace prosecuzione degli studi e per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro. Solo in questo modo si potrà restituire dignità alla formazione conseguita, di cui l'esame di maturità costituisce il coronamento e soltanto l'aspetto finale. L'altro momento altrettanto importante che in Commissione ha marcato le distanze tra maggioranza e opposizione è stato quello relativo alla composizione della commissione Su questo punto occorre rilevare la nostra divergenza con la maggioranza, riaffermando la contrarietà al ritorno ad una composizione mista della commissione d'esame che già in passato si è rivelata inefficace e costosa perché il problema, come ripeto, sta a monte, non a valle, nel senso, cioè, che bisogna restituire valore e serietà all'intero percorso del processo scolastico e non marcare l'accento soltanto sull'ultimo anno. La soluzione per noi ottimale è pertanto quella che prevede che la composizione della commissione rimanga a carattere interno e che solo la figura del presidente sia esterna. E ciò per due motivi: il primo, perché dev'essere rispettosa delle autonomie delle istituzioni scolastiche; in secondo luogo, perché la commissione è impegnata a salvaguardare e a portare a compimento l'interpretazione che le scuole danno al proprio progetto educativo e del quale, a conclusione dell'esame finale, vogliono essere protagoniste attive e non spettatrici passive. Se così è, conseguentemente, il nostro disaccordo permane per intero anche sul vincolo territoriale previsto sulla nomina dei commissari esterni, sul cui operato graverebbe il rischio di condizionamento ambientale a scapito di una maggiore trasparenza e serietà dell'esame. Un discorso a parte va fatto per le prove d'esame. Riteniamo vada superato il ruolo del Ministro che decide su tutto e su tutti, cercando piuttosto di valorizzare gli enti preposti al buon funzionamento della scuola: un valido esempio è l'invalsi il quale, se investito di questo problema, può farsi carico di predisporre le prove d'esame centrandole maggiormente sulle competenze, perché è sulla corrispondenza dei criteri e della certificazione delle competenze che si gioca la qualità d'istruzione del nostro sistema scolastico e il confronto con gli *standard* europei. Il nostro disegno di legge prevede infatti che la terza prova venga predisposta e gestita dall'invalsi. L'Italia è ancora uno dei due Paesi al mondo - l'altro è la Francia - in cui il Ministro sceglie le prove d'esame. Non ce ne rendiamo conto o facciamo finta di nulla. Tutte e tre le prove devono avere degli obiettivi mirati: la prima, quello di accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, dev'essere indirizzata ad accertare le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio; la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, va preparata ed elaborata sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. Noi riteniamo su questo punto, in divergenza con il disegno di legge presentato dal Governo, che i testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta vengano organizzati ed elaborati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione, mentre la terza prova - come ho già detto - dovrebbe essere predisposta e gestita - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 - dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Noi attribuiamo alla terza prova una funzione fondamentale, in primo luogo perché riteniamo che essa vada strutturata in modo tale da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale sia per gli apprendimenti fondamentali sia per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; in secondo luogo, perché essa accerta, oltre ai livelli di padronanza linguistica della lingua inglese, anche quelli della eventuale seconda lingua comunitaria. A conclusione del mio intervento, signor Presidente, sento di poter affermare che il provvedimento che ci accingiamo a varare, pur se concepito e maturato all'interno di un ampio e costruttivo dibattito, necessita, dal nostro punto di vista, di ulteriori miglioramenti. E, in tal senso, gli emendamenti da noi presentati non sono finalizzati ad alcun obiettivo ostruzionistico, ma intendono dare un contributo di proposta e di soluzione a questo importante problema. Ciò nella consapevolezza e responsabilità che un disegno di legge, quando giunge al vaglio dell'Assemblea, si sottopone e si apre sempre a nuovi sguardi, a nuovi perfezionamenti, a sempre più avanzate ottimizzazioni.

spalle una storia tormentata, come il collega Asciutti ed altri - la stessa relatrice - hanno ricordato, sull'esame una volta detto di maturità e ora di Stato, che sta modificando i suoi confini.

che lanciò i quattro pilastri dell'educazione per il 2000: imparare a conoscere, imparare a fare, imparare ad essere

Di qui il primato della centralità delle competenze. Nel 1999 a Bologna era stata appena avviata la riforma Berlinguer quando fu avviato quel processo sottoscritto da 29 Ministri europei dell'istruzione superiore, un processo ancora valido per realizzare entro il 2010 obiettivi comuni a tutta l'Europa: il sistema formativo fondato su due cicli, un sistema comune di crediti didattici, una dimensione europea di tutta l'istruzione superiore, la cooperazione tra gli Stati europei nella valutazione della qualità. Quindi, avvertimmo e avvertì la società italiana che nella società dell'informazione, della diffusione delle nuove tecnologie, della ricerca scientifica non fosse nostro soltanto il compito della valutazione della maturità del singolo studente, ma occorreva dotarlo di conoscenze e competenze chiaramente afferibili a criteri oggettivi e largamente condivisi. Di qui anche, con tutte le sue contraddizioni ed impotenze, la riforma Berlinguer e l'evoluzione dei criteri di valutazione: il sistema dei crediti, la nascita della terza prova (con il suo carattere autonomistico e pluridisciplinare), il ruolo del colloquio e della tesina, e così via. Non ci nascondiamo le difficoltà su cui in Commissione hanno unanimemente riflettuto maggioranza e opposizione; per quello che ho potuto seguire (non sono una specialista), posso valutare una ricerca reale di dialogo, di comprensione, di nuova ricerca, di nuove tesi. Ora, Ora, noi siamo consapevoli che la riforma che proponiamo non è una riforma omnicomprensiva, ma siamo anche consapevoli del fatto che ci siamo trovati di fronte ad un esame ormai svuotato di senso. Questo è stato il nostro problema: un esame ormai svuotato di senso. Con commissioni tutte interne, in fondo era semplicemente, due giorni dopo, il doppione del normale scrutinio; un colloquio sommario (talvolta gli studenti migliori ne risultavano anche mortificati), a cui i docenti davano uno sguardo distratto. Quindi un esame svuotato di senso e dati che ci preoccupavano ed impressionavano. Abbiamo ascoltato con molta attenzione le riflessioni dei senatori Asciutti e Valditara sul ruolo delle paritarie. Nelle stesse audizioni ricordo di aver sentito rappresentanti di scuole paritarie sommamente preoccupati di rinnovare la serietà dell'esame; talvolta erano rappresentanti di scuole paritarie religiose. Ma noi siamo di fronte a questo dato: nel 2001 i candidati privatisti delle scuole paritarie erano 348, nel 2004, tre anni dopo, erano 19.040 (ecco il costituirsi dei diplomifici), mentre i candidati privatisti nelle scuole statali diminuivano da 28.065 a 22.258. Nelle paritarie noi segnammo una vera e propria impennata verso l'alto delle votazioni e un abuso - diciamo così degli ottisti. Questa è diventata consapevolezza comune, ma questo è il risultato dal 2001 al 2004. Ecco che, negli anni 2005-2006, era nostro dovere svoltare. Diciamo la verità: la deprivazione di senso di questo esame era diventata tale che noi ci siamo trovati di fronte ad un bivio. O si sceglie il modello svedese, statunitense e di alcuni Stati del Canada, per cui, così com'è, questo esame può essere sostituito da un solo più razionale scrutinio generale, alla fine del quinquennio, e decade il valore legale del titolo di studio; oppure si pensa di mantenere a questo esame una sua funzione certificativa di diploma di secondo livello e conclusiva del ciclo di istruzione, e allora bisogna restituirgli serietà. Non dico la serietà che ha il baccalaureato francese, dove, nell'anonimato dello studente, migliaia di docenti e correttori esterni valutano le prove secondo rigidi parametri, senza neppure sapere a chi appartengono (questo è il modello del baccalaureato francese); ma, con realismo, ritroviamo insieme, di fronte a quel livello di degrado, una nostra ricerca di efficacia, di qualità certificativa e di serietà. Insomma, io credo che tutti, non importa se di destra o di sinistra, dobbiamo ribellarci a questa maturità senza qualità e quindi dare a questo provvedimento tanto atteso qualche significativa risposta. Noi riteniamo di aver dato qualche significativa risposta. Sappiamo che i problemi sono a monte,

Forse questo provvedimento non è sufficiente: è un tetto nuovo in un edificio che ha ancora molte crepe,

penso alla riflessione avanzata da «Il Sole 24 ORE», che guardava con attenzione al nostro percorso, al nostro comune percorso - che pensava che ce l'avremmo fatta. Nessuno, proprio nessuno. Ma ecco che questo vecchio modello, che così vistosamente mostra le sue insufficienze, ora viene corretto nei punti fondamentali, riguardanti l'ammissione all'esame di Stato, l'obbligo di aver saldato i debiti formativi, il rigore per i privatisti, l'esame preliminare per i candidati esterni,

non a ciò che faremo nel momento in cui lo voteremo, ma a ciò che delegheremo il Governo a fare. Chiamo l'articolo 2 di questo provvedimento un vero e proprio percorso dell'eccellenza:

a tutela di un percorso di eccellenza per gli allievi migliori è o non è spazio del nostro futuro? Noi non abbiamo riformato la scuola superiore, ma abbiamo provato a reagire ad un percorso di

l'intervento del collega Asciutti, mio Capogruppo in Commissione, ha già dato un segnale chiaro dell'atteggiamento di Forza Italia rispetto a questo disegno di legge. Tra l'altro, è il primo disegno di legge del ministro Fioroni ed è la carta di presentazione del Dicastero retto dal nuovo Ministro. È la prima azione concreta del Governo Prodi in un settore delicatissimo come quello della scuola

lo abbiamo ascoltato, seguito anche con un certo *pathos* nelle maratone volte ad inseguire i finanziamenti, prima tagliati, poi forse restituiti: staremo a vedere in finanziaria, alla fine, se questi se questi passaggi da una stanza all'altra dei componenti del Governo riusciranno davvero a salvare qualcosa, dal punto di vista finanziario, per la nostra scuola. Lo abbiamo anche seguito nelle vicende che riguardano i precari della scuola; non lo sappiamo ancora, ma capiremo se i precari potranno diventare insegnanti di ruolo oppure no; quali saranno i programmi. Ma la relatrice, senatrice Soliani, oggi ci consiglia

legislatura per conoscere quale sarà la suddivisione delle stanze della casa dove i nostri studenti si formano per la vita,

quali le piccole soppressioni o quali gli aiuti alla comprensione di precedenti norme, ho l'impressione che dovremo attendere molto. Persino la visione crociana che ci viene offerta oggi - penso con simpatia ai colleghi della sinistra estrema - il dover cioè essere tutti quanti ricondotti, per bocca della relatrice di centro-sinistra, senatrice Soliani, alla idea crociana della scuola deve essere un esercizio piuttosto forte per voi! Ma tanti auguri! Se Croce serve a specificare o a far digerire un qualunque disegno di legge, ci sta bene. Per noi Croce non è certo uno scandalo nella conversazione generale.

ben chiaro in testa qual è il progetto complessivo cui si tende e quale il risultato finale cui si ambisce, quali sono i passaggi o le prospettive. Allora, mentre seguiamo l'andamento veloce da maratoneta del nostro Ministro alla rincorsa di fondi e quello delle sue discussioni con i sindacati per quanto riguarda le questioni pregnanti del precariato, a noi non resta che che la valutazione che oggi rende la senatrice Negri e che prima di lei la senatrice Carloni hanno voluto rassegnare a questo dibattito parlamentare.

siete andati a scomodare una serie di argomentazioni per cui vi dico sin da subito che siamo assolutamente d'accordo! Non cercate disunione, laddove non c'è perché non ha motivo di essere.

i professori quale bene strumentale alla formazione dei nostri giovani, dei giovani italiani del futuro? Chi, senatrice Carloni, non ritiene che il Sud ha nella scuola un momento di riscatto e di promozione sociale?

luogo dove si misurano con il mezzo punto, con il credito formativo alla virgola, la capacità e l'inventiva del giovane.

ha sottolineato che, rispetto a condizioni eguali, di cittadini ed insegnanti eguali, perché eguali sono le abilitazioni conseguite, lo Stato laico non può porsi problemi di diversità, non può porre diversità di atteggiamento.

L'obiettivo dello Stato è, innanzi tutto, quello di dare una formazione culturale e quindi scolastica al maggior numero di cittadini possibile e,

è il vicino che abbiamo in casa, che concorre con noi, con gli stessi diritti e potenzialità dei nostri figli e dei nostri giovani, ad occupare tutti gli spazi di governo dell'Europa. Se i nostri giovani non saranno attrezzati ad occupare questi spazi di governo, perché fin dalla formazione scolastica non hanno le medesime potenzialità

Allo Stato non deve interessare se quella formazione di eccellenza viene data da un'istituzione pubblica o privata: allo Stato deve interessare che arrivi la formazione di eccellenza.

ad un'antica triremi greca, con tre file di vogatori sulla fiancata destra e tre file di vogatori sulla fiancata sinistra molto scarsamente sincronizzati;

Se il Governo non avrà il coraggio di dire alla propria maggioranza, eterogenea che sia, che bisogna fare delle riforme per mettere i nostri giovani ed il nostro sistema Paese in condizioni di essere competitivi con il sistema Europa, e quella della scuola è una di queste riforme,

bisogna dare in pasto ai propri *supporter* elettorali messaggi importanti di incoraggiamento, ma che alla fine c'è un Governo che deve prendere delle decisioni

che riguarda il mondo della scuola ma, ancora una volta, oggi ascolto un intervento anacronistico sulla questione della terza prova. Oggi desideriamo fortemente, lo dico come Gruppo di Forza Italia, interloquire con il mondo esterno, con la scuola, con i discenti, con gli insegnanti e tutto il mondo del sindacato. Vogliamo discutere con il mondo della scuola pubblica e privata,

la sfida è veramente molto più sottile. Oggi c'è un Sud-Est asiatico che si affaccia alle nostro frontiere mediterranee, non più alle nostre frontiere mitteleuropee. Oggi la cultura si compone anche di tutta una serie di arricchimenti - per qualcuno potranno essere depapeuramenti - della nostra cultura nazionale che provengono da nuovi confini. Rispetto a tali nuovi confini,

La Sicilia o la mia Ragusa possono o debbono per forza avere una diversità di sensibilità ma anche di missione, dal punto di vista dell'azione dello Stato, rispetto a Sondrio, a Trieste, a Genova o a quant'altro. È chiaro che è La scuola viva è la scuola che si incarna, e non è nozionismo, non è solo dottrina: la scuola è vita, la scuola è preparazione. Infatti la viviamo in quella fase, dai sei ai diciotto anni, dopo

il sei, la sufficienza in tutte le materie, la terza prova specifica: viviamo come un momento di altissima burocrazia sarebbe necessaria anche la creatività, che è uno degli aspetti fondamentali dell'essere giovani, dell'essere una nuova generazione: si dice nuova generazione proprio perché innova un sistema sociale che

Se siamo punitivi e basta soltanto al momento dell'esame, sembreremo ingiusti, sembreremo repressivi. Se siamo punitivi e basta al momento degli esami, senza essere riusciti a dare tutte quelle dotazioni delle quali è assolutamente necessario sia fornito il giovane moderno, il giovane del terzo millennio, per competere e nella società e nel mercato rispetto agli altri giovani del pianeta, è chiaro che tutto apparirà estremamente estremamente chiuso, tutto estremamente rigido, estremamente punitivo: non sarà la scuola che ti accompagna ma la scuola che ti bacchetta. E allora, per concludere signor Presidente, signor Ministro, questo le chiediamo:

ci dia la possibilità di discutere di disegni strategici del Dicastero da lei presieduto; ci dia la possibilità che, sugli indirizzi generali, ci si possa anche scontrare, ci si possa anche diversificare nelle posizioni,

Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, la decisione del Governo di mettere all'ordine del giorno la modifica degli esami di Stato noi l'abbiamo salutata con soddisfazione: una decisione giusta, un provvedimento necessario e urgente. A sottolineare tale urgenza stanno molti segnali e molte ragioni. Innanzitutto l'esigenza di contrastare con determinazione il dilatarsi della piaga dei diplomifici, la perdita reale del valore dei titoli di studio, il canto suadente di molte sirene che vorrebbero addirittura mettere in discussione il valore legale di questi titoli, una università che sempre meno tiene conto dei risultati conseguiti negli esami di maturità dalle proprie matricole. Tutte le componenti della scuola, come dimostrano le audizioni tenute presso la 7a Commissione di questo ramo del Parlamento, ci hanno rafforzato nel convincimento che la riforma degli esami varata nel 2001 su proposta del Governo allora in carica avesse fatto del male, molto male alla scuola. Urgenza significa anche che siamo chiamati ad assumere un provvedimento entro scadenze tali che permettano l'effettuazione dell'esame di Stato, caratterizzato dalle nuove regole, già al termine dell'anno scolastico in corso. Esiste un'attesa generalizzata in questo senso e se il Parlamento non dovesse corrispondere a queste aspettative, reale diventerebbe il rischio di una ulteriore dequalificazione dell'esame di Stato e di un ulteriore danno al sistema scolastico. Che la normativa in vigore dal 2001 non fosse convincente non stava solo nella nostra riflessione: anche i senatori dell'opposizione, con la presentazione di loro proposte di riforma, confermavano necessità e urgenza di cambiamento. Non vogliamo qui evidenziare le diversità dell'impianto delle proposte presentato dai colleghi di Forza Italia rispetto a quelle di Alleanza Nazionale, evidente per altro nella parte relativa alla composizione della commissione di esame, ma cogliere come l'urgenza di una riforma fosse tema vasto e trasversale anche nell'emiciclo di quest'Aula. Con i cambiamenti introdotti nel 2001, nel contesto della legge finanziaria, senza un dibattito specifico, non fu attuata una riforma, ma un taglio delle commissioni di esame, che da allora sono composte tutte da commissari interni. L'impianto dell'esame di Stato costruito con la legge del 1997 rimase invariato, ma le modifiche apportate alla composizione delle commissioni hanno comportato conseguenze molto negative. Esse furono presentate come una soluzione facilitante per gli studenti, ma gli studenti italiani non hanno bisogno di simili facilitazioni: hanno bisogno di una preparazione seria e qualificata e di un titolo di studio che conseguentemente possa essere speso nel mercato del lavoro e della formazione. Questo di oggi è un primo importante atto della politica scolastica del centro-sinistra, una politica che si integra con passaggi importanti che affronteremo nelle prossime settimane, primo fra tutti il tema cruciale dell'innalzamento dell'obbligo. Proprio perché è il primo atto, crediamo sia utile, in occasione di questa discussione, non solo sugli aspetti di merito della proposta di riforma dell'esame di maturità, ma anche sui valori e sulle aspirazioni che con questo atto di riforma vogliamo dichiarare e porre all'esame del Paese. il primo punto è la nostra chiara volontà di ridare valore e serietà al nostro sistema scolastico. Credo che dobbiamo partire da qui, senza scomodare le statistiche, che pure hanno qualche valore; se empiricamente osservassimo i risultati degli esami di ammissione all'università da parte dei nostri studenti, coglieremmo alcune difficoltà del sistema scolastico, indeciso a tutt'oggi tra una funzione specialistica ed un'altra generalista, mai pienamente definita, e coglieremmo quanto dannoso sia stato eliminare quei necessari riti di passaggio all'età adulta, capaci di mettere i nostri giovani nella necessità di misurarsi con il grande tema dell'ingresso nell'età adulta della maturità. Per questo riteniamo che la linea guida debba essere quella di un esame di Stato equo e rigoroso e credo che il lavoro della 7a Commissione ci consegni il risultato più equilibrato possibile, un equilibrio che ha tenuto conto delle aspettative tanto del corpo insegnante, quanto del mondo studentesco. Se questo era, all'inizio dei lavori, l'obiettivo della riforma, ne abbiamo tratto le giuste conseguenze, anche nella definizione della norma. La soluzione della commissione mista è quella che maggiormente garantisce un punto di equilibrio tra la necessità di un giudizio terzo e la continuità con il percorso scolastico compiuto nelle scuole dell'autonomia che, attraverso i piani di offerta formativa, declinano i *curricula*. Per questo faccio riferimento alla categoria dell'equilibrio: equilibrio tra la necessità di un giudizio omogeneo su tutto il territorio nazionale, elemento necessario a garantire il valore legale e sostanziale del titolo di studio, per noi imprescindibile, e la necessità di valorizzare un contesto come quello delle scuole autonome. L'autonomia scolastica non è un bene da riscoprire quando si tratta di scaricare difficoltà sulle scuole, ma è ormai un tratto costituivo, fondante, del nostro sistema scolastico. Il provvedimento del Governo, finalmente, affronta la grande questione dell'orientamento, questione troppo spesso disattesa nel nostro Paese e al centro, invece, delle politiche di molti Stati europei. Su questo terreno non possiamo non sottolineare l'ambizione della delega che il provvedimento affida al Governo. Essa tenta di raccordare il mondo della scuola e dell'università in un disegno coerente. Crediamo però che la coerenza del disegno sarebbe stata rafforzata dall'identificazione degli opportuni strumenti di orientamento e raccordo anche con il mondo del lavoro, per un ingresso consapevole dei giovani nell'attività professionale, visto che il nostro sistema scolastico si compone di diversi percorsi, tutti di pari dignità, il cui esito non è sempre l'ingresso all'università. La complessità introdotta nella nostra Costituzione dall'articolo 117 non ci ha consentito di affrontare esaurientemente la questione, ma spero che, in sede di Conferenza unificata prima e di iniziativa parlamentare poi, il Governo sappia affrontare anche questa grande sfida. L'allargamento dell'orientamento agli istituti di formazione tecnica superiore e la valorizzazione della formazione scientifica, proposte che abbiamo condiviso con la Commissione, già indicano questa sfida futura di un nuovo raccordo, al termine della secondaria e non prima, con il lavoro e la formazione lungo il corso della vita. Sono primi segnali che dovremo approfondire, anche per i grandi effetti che avranno sul Paese e sulle competenze dei nostri ragazzi. Com'è noto, il nostro sistema universitario non riesce a soddisfare, soprattutto nell'area scientifica, la domanda di personale qualificato che proviene dal sistema delle imprese, con un'incidenza negativa sulla competitività del Paese. Insomma, dopo questo primo passo altri passi dovremo rapidamente percorrere, restando saldi come oggi sui princìpi e sul programma, come ad esempio la centralità del valore legale del titolo di studio, confermata e rafforzata dal provvedimento in esame. Nel quadro della riforma del secondo ciclo della legge Moratti (fortunatamente sospesa) si prefigurava per l'appunto un quadro per cui il diploma sarebbe stato sostituito da una certificazione per l'accesso all'università, precluso al settore dell'istruzione tecnica e professionale. Si trattava di un quadro utile a perpetuare e accentuare un male endemico del sistema scolastico italiano, evidenziato anche da recenti studi sociologici: la staticità sociale per cui, nonostante la liberalizzazione degli accessi, l'istruzione universitaria e, in seguito, le carriere, sono riservate ai figli di genitori con titolo di studio e situazione sociale e culturale elevata. Nel programma di Governo dell'Unione non ci si limita certo a prendere atto di questa situazione ingiusta e dannosa per il Paese. Non si propongono pertanto aggiustamenti tecnici ma una riforma, a cominciare dall'elevamento dell'obbligo scolastico che modifichi questa staticità staticità sociale, che imprima, per quanto può fare la scuola (e può far molto), un rilancio dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

ad un ragionamento, ad una discussione, ad un'analisi che certo meriterebbero un approfondimento ed un aggiornamento, ma lo fa partendo dalla parte sbagliata:

offendendo la classe degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Non penso non ci fosse serietà.

strilli e dolori, come è naturale, ma se una riforma non lacera degli interessi acquisiti è una riforma che non lascia traccia. Non mi pare che dobbiamo partire da qui. Eppure, da allora poi l'esame di Stato

siamo sicuri che con questa riforma, con le commissioni miste, con l'esame preventivo di ammissione non ci sarà più autoreferenzialità?

Stato. Il coraggio poteva essere quello di interagire con l'università e con il mondo delle professioni per distinguere,